Comunico che in data 23 novembre 2020 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:* «Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154,

lavori». Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito il calendario dei lavori fino al 2 dicembre. L'ordine del giorno della seduta odierna prevede la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge concernente statistiche in tema di violenza di genere. Nella seduta di domani, alle ore 9,30, avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri della difesa, dell'istruzione e per gli affari europei. Alle ore 13 sarà discussa la Relazione al Parlamento sull'autorizzazione al piano di rientro verso l'Obiettivo di medio periodo, per la cui approvazione è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. La settimana dal 30 novembre al 4 dicembre sarà prevalentemente riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al decreto-legge ristori. L'Assemblea si riunirà mercoledì 2 dicembre, alle ore 9,30, per comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Il calendario potrà essere integrato con l'esame del rendiconto e del bilancio interno del Senato. Su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze di riferire alle Camere in vista della riunione dell'Eurogruppo del prossimo 30 novembre sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità e l'introduzione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico, è stato stabilito che tale informativa abbia luogo presso le Commissioni competenti.

Non nascondetevi dietro alla Commissione o a qualcos'altro. Domani - ed è l'invito che rivolgo - c'è tutta la possibilità per discutere di questo tema.

sì alla Commissione, ma anche all'Assemblea! Il Parlamento è Commissioni e Aula.

Forse c'è il timore che si dia troppo peso a questa riforma o riformetta, alla pillola addolcita che si vuole dare al MoVimento 5 Stelle per poi obbligarlo ad aderire al MES? Signori, c'è una grande opportunità

10,45 saranno sicuramente finite. Non vediamo ragioni per aspettare le ore 13 - e anche per ragioni logistiche, in quanto sappiamo quanto sia difficile spostarsi in Italia in questo periodo

ma anche in Assemblea. L'argomento è estremamente importante, coinvolge di sicuro tutti i settori del Paese e non può essere confinato nel pur prestigioso e altamente rispettato

interventi più che legittimi dei membri della maggioranza, ma che di fatto nascondevano l'imbarazzo nel voler portare in Assemblea la discussione. Come ha già detto il capogruppo Romeo, noi non ci nascondiamo. Il MES è sicuramente un argomento su

argomenti che riguardano la Nazione e gli indirizzi che questo Governo dovrà avere all'interno della Commissione europea e dell'Eurogruppo.

Presidente, credo che questa discussione sul calendario dei lavori sia importante, perché sta nascondendo un non detto che io invece vorrei esprimere fino in fondo. fondo. Se uno ascoltasse soltanto le parole del senatore Romeo, si chiederebbe per quale ragione la maggioranza non accorda

la discussione non verte sull'utilizzo o meno del MES, ma sulla riforma del MES, che è un'altra storia rispetto alla questione su cui maggioranza e opposizione si sono divise e si dividono al loro interno. Il problema è un altro, signor Presidente. Qui c'è una forza politica - lo dico soprattutto a Forza Italia e a Fratelli d'Italia - che sta sistematicamente lavorando per interrompere ogni forma di dialogo fra maggioranza e e per impedire di discutere di qualunque provvedimento che riguarda il Paese e l'emergenza sanitaria ed economica in cui si è cacciato. Questa forza politica è la Lega. Lo dico perché è dalla Conferenza dei Capigruppo di ieri che la Lega e Massimiliano Romeo, in particolare, cercano il pretesto per interrompere ogni discussione che ci veda lavorare insieme. Romeo ha abbandonato la Conferenza dei Capigruppo quando ancora i senatori Capigruppo della maggioranza stavano intervenendo. Non ha dato la possibilità di fare nemmeno una proposta,

alla Conferenza dei Capigruppo - lo dico a Forza Italia e a Fratelli d'Italia - sa benissimo che le forze politiche di maggioranza hanno dato disponibilità per la seduta d'Assemblea, per

gli viene l'allergia: il tema è questo. Egli ci impedisce di dialogare e impedisce alle forze parlamentari di svolgere un percorso unitario in un momento in cui l'unità delle forze politiche dovrebbe dovrebbe essere prioritaria. *(Commenti)*. Chiedo a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, che sono testimoni del fatto che il senatore Romeo ha abbandonato la Conferenza dei Capigruppo, di non assecondarlo.

le proposte che venivano dalla maggioranza! Pertanto, signor Presidente, ristabiliamo la verità. A noi interessa il dialogo. Interesserebbe, da ieri, votare insieme almeno il calendario. In quest'Aula non si riesce neanche a votare insieme il calendario, perché il senatore Romeo e la Lega ce lo impediscono. È ridicolo!

di dire altro rispetto a quanto la Lega, strumentalmente, mette in campo.

La prima proposta, pur di non votare il calendario insieme alla maggioranza, pur di distinguersi, pur di boicottare il forte forte tentativo di confronto che stiamo portando avanti, è stata quella relativa alla data della presenza in Senato del ministro Speranza. Noi abbiamo chiesto, come Parlamento, proprio per svolgere un ruolo centrale anche sui DPCM, che il Governo ci venga sempre ad aggiornare e a informare. Tant'è che il ministro Speranza ha avanzato esattamente la proposta di venire in il senatore Romeo ha una questione rilevantissima: lo vorrebbe fare ventiquattr'ore prima, pur di votare contro il calendario. In aggiunta a questo, il ministro Speranza, viste le continue accuse di alcuni mezzi di comunicazione e anche di alcuni partiti politici sulla preparazione del Governo e del nostro sistema sanitario, verrà a comunicarci il piano di vaccinazione, che è pronto che è pronto perché si dovrà realizzare fra poche settimane. Quindi, quella presenza è importantissima per il Parlamento, per il Senato della Repubblica. Andare a cavillare sui tempi, prima o dopo, senza centrare l'importanza di quel passaggio parlamentare, testimonia un arroccamento su posizioni che tendono a boicottare ed escludere un confronto serio e collaborativo in una situazione di emergenza per il nostro Paese. Aggiungo, sulla questione della disponibilità del ministro Gualtieri, che oggi ho sentito il senatore Romeo assurgere a difensore

per fare un confronto. È già previsto un voto. Signor Presidente, su questi temi è previsto un voto, che è già stato calendarizzato. Il 9 dicembre verrà qui in Aula il presidente Conte, prima del Consiglio d'Europa,

deve creare dei presupposti, deve creare consenso, deve servire a dare una linea di comportamento del nostro Governo, è certo che deve essere svolto in Commissione e non - come è stato chiesto stamani stamani - in Aula, magari con interventi di cinque minuti. Noi vogliamo una cosa seria. Vogliamo parlare con franchezza e determinazione sul futuro del nostro Paese. Vogliamo avere la possibilità di approfondire i temi. Non c'è bisogno di utilizzare l'Aula

di dialogo. Credo che sia giunto davvero il momento di fare un passo in avanti e di dimostrare al Paese che l'attuale classe politica - quindi tutti noi - è in grado di gestire questa emergenza, di dare concretezza alla volontà di dialogo e di votare un calendario di buonsenso, che prevede il coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni del Governo, che sono importanti per il nostro futuro.*(Applausi)*.

è un po' avvilente che si debba venire in Aula a discutere di cose che forse, se si avesse la volontà di sentirsi e di ascoltarsi, parrebbero a tutti di buonsenso.

fatto che l'Italia si presenti all'Ecofin sempre con dibattiti che onestamente rischiano di essere fuorvianti: siamo l'unico Paese in Europa che discute dalla mattina alla sera,

con un dibattito in Aula, che rischia di essere solo propagandistico, il nostro Paese si presenti all'Ecofin con una discussione assolutamente sfilacciata e nessun tipo di approfondimento. È arrivato il momento di dare una prova di serietà.

a fare una discussione, ma credo che, se siamo delle persone serie, dobbiamo assumerci la responsabilità una volta per tutte davanti al Paese: dobbiamo fare una discussione seria e tecnica per poter davvero provare a entrare nel merito, e non rinfacciarci le cose gli uni con gli altri in dibattiti che rischiano di essere inutili e ideologici. Signor Presidente, penso ancora che sia assolutamente utile che l'informativa venga svolta all'interno delle Commissioni e lei ovviamente deciderà, come Presidente, a quale Commissioni affidarla.

potete benissimo votare contro la proposta avanzata dalla Lega. Ma Forza Italia e Fratelli d'Italia, ai quali in questa occasione avete cercato un po' di strizzare l'occhiolino per cercare di dividerli, hanno fatto una proposta analoga. Quindi, votate contro la proposta della Lega, ma votate a favore della proposta di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, che dice la stessa cosa. Così almeno non sarà la Lega che, abbandonando la Conferenza dei Capigruppo, condiziona il Parlamento. Sarete voi, con il voto che fra pochi minuti darete, a stabilire se avete il coraggio come maggioranza di venire ad affrontare il tema del MES, perché non avete paura di andare davanti agli italiani e di far vedere come la pensate. Questa è la strada giusta che dovete mettere in evidenza. *(Applausi).* È il vostro voto che determina le scelte. C'è una proposta per lunedì, giusto? Saremmo entro il 30 novembre, ossia il termine stabilito dal ministro Gualtieri, e ci sarebbe tutto il tempo per preparare assolutamente l'Assemblea.

non c'è alcun tipo di modifica del calendario per noi. Noi voteremo la proposta che ha fatto Forza Italia, ossia che il ministro Gualtieri venga lunedì in Aula a mezzogiorno. Così, tolte le nostre proposte, non ci sono più scuse, signori. Avanti, forza, coraggio. Tirate fuori

proprio per agevolare il computo dei voti, attese alcune riserve che sono state espresse in votazioni precedenti. Naturalmente, questa votazione elettronica sarà senza indicazione dei nomi.

qualche giorno fa il Presidente della Commissione bicamerale antimafia ha rilasciato dichiarazioni sgradevoli nei confronti dei cittadini calabresi, dei malati oncologici e della compianta collega Santelli. Abbiamo chiesto, come si deve fare in questi casi, che vi fossero delle scuse perché è possibile a chiunque incorrere in un infortunio o in uno scivolone. Il presidente Morra, anziché scusarsi, ha rilanciato con dichiarazioni ancora più antipatiche e inopportune. Abbiamo letto una serie di prese di posizione di tutti gli esponenti istituzionali di maggioranza e di opposizione che si univano alla nostra richiesta di scuse che, a questo punto, signor Presidente, non credo possano più bastare. possano più bastare. Abbiamo comunicato, pertanto, formalmente per iscritto che non parteciperemo più alle riunioni della Commissione bicamerale antimafia e dei suoi Comitati fino a quando la questione non sarà chiarita nei modi e nei tempi opportuni. Chiediamo di sapere cosa intenda fare la maggioranza sulla vicenda: ci dica se ritiene che una Commissione bicamerale di garanzia così importante debba proseguire i suoi lavori senza l'opposizione (e in questo caso ne prenderemo atto) o se invece ritiene di

Signor Presidente, per riprendere l'intervento del collega Vitali, voglio citare una dichiarazione che mi è stata sottoposta pochi secondi fa: «Morra non avrebbe dovuto dire quella frase»; l'ha pronunciata poco fa il procuratore capo di Catanzaro Gratteri dicendo, tra l'altro, che tra le mille intercettazioni telefoniche che ha letto durante la sua attività di magistrato non ha mai trovato il nome di Jole Santelli, né come soggetto di intercettazioni, né come persona tirata in ballo da altri delinquenti o presunti delinquenti. scritta una brutta pagina in queste ore e onestamente questo intervento avrei voluto evitarlo. C'è stato un crescendo perché, con quella frase pronunciata dal senatore Morra è stata attaccata una persona che oggi non c'è più e alla quale mandiamo da questa Aula un caloroso abbraccio soprattutto in una giornata come questa.

Presidente, sono stati inoltre attaccati tutti i malati oncologici, persone straordinarie che devono vivere intensamente la loro vita e che hanno da trasmetterci valori indelebili di cui tutti dovremmo essere portatori. (*Applausi*). Sono poi stati offesi tutti i calabresi per una scelta libera e democratica che hanno fatto soltanto

in passato sulla sanità lucana.

ma il vessillo dell'antimafia non lo lasciamo, né al senatore Morra, né al MoVimento 5 Stelle, perché quel vessillo è di tutti gli italiani, della stragrande maggioranza degli italiani onesti. È chiaro che noi continueremo a non partecipare ai lavori della Commissione, Presidente. È chiaro perché il ruolo di garanzia della Presidenza della Commissione antimafia, che richiede equilibrio e senso di responsabilità, così come è interpretato adesso finisce per delegittimare tutta la Commissione antimafia. *(Applausi)*. E soprattutto, Presidente, fino ad oggi

ha superato qualsiasi limite, qualsiasi tipo di decenza. Mi rivolgo alle forze di maggioranza: tanti esponenti della maggioranza hanno stigmatizzato le frasi del presidente Morra. Carissimi colleghi di maggioranza, abbiate uno scatto di orgoglio e di dignità, perché tocca a voi e non a noi chiedere le dimissioni del presidente Morra! *(Applausi)*. Pronunciate questa parola, abbiate uno scatto di orgoglio e di dignità!

Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia, nelle persone del sottoscritto quale Capogruppo del partito in Commissione antimafia, insieme al senatore Ciriani e alla deputata Ferro, si è visto costretto a comunicarle, nella giornata di sabato, che non avremmo più preso parte alle sedute della Commissione perché, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, le dichiarazioni del presidente Morra sono indegne dell'alto livello istituzionale che ricopre. Presidente, a noi oggi dispiace ancor di più, dopo le cose gravissime che abbiamo già registrato, vedere il presidente Morra rimanere seduto nel momento in cui in quest'Aula viene evocato ancora una volta il nome di Jole Santelli *(Applausi),* un presidente di Regione eletto liberamente dai calabresi, ma soprattutto - mi sia consentito dirlo - una donna che nel momento in cui era a rischio la sua vita sentiva ancora di essere impegnata per la propria gente e per amore della propria terra. Non si possono lanciare pietre, non si possono adombrare meschine quando siamo al cospetto di persone che andrebbero soltanto elogiate e prese come esempio. Non capiamo, presidente Morra, per quale motivo un malato oncologico non possa essere votato da un cittadino. Siamo tutti sotto al cielo; i malati oncologici possono guarire. Qual è è la logica della sua dichiarazione? È assolutamente incomprensibile e fuori luogo, così come non si capisce quale sia l'incapacità del popolo calabrese nello scegliersi i propri rappresentanti. Mi sembra che alle elezioni politiche del 2018 i calabresi, come gran parte del popolo meridionale, hanno votato per i 5 Stelle in maniera massiccia. In quell'occasione, allora, i calabresi e i meridionali erano persone in grado di scegliere e di scegliere il meglio *(Applausi)* mentre oggi sono incapaci di intendere e di volere e completamente piegati alla logica dei corrotti e dei malavitosi? Nessuno ha la patente di onestà che può conferire agli altri e offende ancor di più quello che abbiamo ascoltato nelle ore successive, quando ci siamo sentiti dire che era in atto un complotto che voleva Morra fuori dalla Commissione antimafia per fare il gioco di forze oscure. È un'accusa che noi di Fratelli d'Italia rifiutiamo nella maniera più completa, e lo testimonia la nostra storia da sempre schierata per la legalità e per lo Stato che tutti rappresentiamo. il vessillo esclusivo della lotta alla malavita e alla corruzione. Presidente, le chiediamo un intervento forte e autorevole, come lei è in grado di fare, per fare chiarezza su questa vicenda,

presidente Morra, che alle spalle di determinate decisioni e della sua esclusione non ci sia una parte politica molto diversa dall'opposizione. *(Applausi)*.

ringraziare, tra le tante persone, una cittadina di Padova, che qualche sera fa mi ha espresso la sua opinione su questa vicenda. «Cosa guardo per capire se un politico è autentico? Non quando dice la cosa più comoda, la più ovvia o porta acqua al suo mulino ma quando ha il coraggio di dire ciò che altri tacciono, anche se gli nuocerà».

sospendo la seduta. Non create assembramenti, uscite. Mi pare che si stia trattando un tema molto delicato e vorrei che ci fosse silenzio.

intervento. Capisco che alla Lega dia fastidio l'opinione di una cittadina, ma ho riportato parole che non sono mie. Ho riportato parole che mi vengono dalla gente e questo evidentemente dà fastidio, perché la lingua batte - soprattutto quella del popolo - dove il dente duole. questa signora mi ha detto che non guarda se una persona fa la cosa più comoda, o che le fa più comodo, ma quando ha il coraggio di andare controcorrente, a maggior ragione se sa riconoscere un errore proprio. Il presidente Morra si è scusato per quella parte delle sue parole che sono andate oltre il suo spirito e le sue intenzioni, soprattutto nel passaggio magari dal verbale alla trascrizione stampata e ciò, all'occhio di questa signora, lo rende credibile. Mi ha detto di aver ascoltato le sue parole e di aver ascoltato quelle che vengono anche dalle altre forze politiche e le loro reazioni e di essersi fatta una sua idea: non sta dando una dimostrazione di credibilità un certo centrodestra tracotante, muscolare spregiudicato, che prima ha scelto una figura di alto profilo istituzionale come Jole Santelli,

una persona che invece doveva rispondere di diversi episodi di corruzione. Qual è la coerenza tra votare all'unanimità in Commissione bicamerale antimafia le linee guida del codice di autoregolamentazione per i partiti nella composizione delle liste

Non si può parlare neanche di un assente, figuriamoci di una persona che è morta. Non si può! Non si può e non si deve! C'è un codice deontologico di comportamento e di condotta oltre il quale non si può andare. Non è possibile. Non si parla di una persona defunta. Non si può infangare il nome di Jole Santelli. Guardi, Presidente, che io di Jole Santelli ho detto il contrario: o lei allora non mi ascolta, oppure già era preparata a censurare le mie parole, lei che dovrebbe garantire il dibattito. *(Applausi)*. Non ho offeso nessuno. Ho detto che era una figura di alto profilo istituzionale e apprezzata in sede di Commissione bicamerale antimafia. Dunque, facciamo uno sforzo per capire le parole, perché altrimenti non ne usciamo. Non si permetta, perché sennò la mando fuori, ha capito? Non si permetta, nei confronti della Presidenza. Abbia rispetto delle istituzioni. Qui manca il rispetto istituzionale

La violenza verbale non ha nulla a che fare con il confronto democratico!

perché se dal centrodestra, almeno la parte più libera e liberale, che oggi si è espressa con toni senz'altro diversi rispetto ad altri e che forse si sta smarcando da un abbraccio un po' un po' ruvido e poco conciliabile con il dialogo politico, se almeno da queste forze non arriva una spiegazione di quel che è successo il cittadino le spiegazioni le deve trovare da sé

La Lega dovrebbe avere il coraggio di dire se i sentimenti buoni e giusti possono essere distorti etichettati come buonismo e dipinti come un male quando si parla di profughi, immigrati e - perché no? - anche di immigrati irregolari. Ho parlato infatti di sentimenti buoni e giusti, basati sulla giustizia, non ideologici e astratti. Mi chiedo perché in questo caso il buonismo è un male e diventa invece una virtù, quando giustamente si difende la dignità della malattia e della morte. Questo è anche stato fatto e non si può negare che su questo ci sia stato un problema, ma non si può fare per nascondere una vergogna inaccettabile... Non si può fare per nascondere una vergogna, inaccettabile e voluta, come porre Tallini in lista e premiarlo poi con la presidenza del Consiglio regionale. Non una parola è venuta dalla Lega su questo. Chi ha speculato allora sul ruolo importante di Jole Santelli? Lega il coraggio di dirlo oggi che su Tallini sono giunti non sospetti, ma accuse gravissime, che lo hanno portato all'arresto per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico-mafioso. Voglio dirlo in questa sede: secondo l'accusa, i rapporti di Domenico Tallini con la cosca Grande Aracri, di Nicolino Grande Aracri, oggi recluso al 41-*bis* nel carcere di Opera, avrebbero riguardato la costituzione di una società, con base a Catanzaro.

una società finalizzata alla distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali, mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie: venti in Calabria, due in Puglia e una in Emilia-Romagna.

fare: ha preso le distanze da quelle parole e solo da quelle, perché molti cittadini si riconoscono nel resto del messaggio, nella sua parte centrale e portante: una trave per un cambiamento che gli onesti di tutta Italia vedono intoccabile e cristallina. La politica in Calabria è deviata dalla 'ndrangheta. *(Applausi)*. La Regione Calabria ha un disavanzo ormai non più sanabile autonomamente; la gran parte di questo disavanzo è dovuto alla gestione della sanità. La Regione Calabria non sta garantendo ai calabresi il diritto alla salute.

Domenico Tallini doveva rispondere per più episodi di corruzione, ma è stato inserito nelle liste e poi premiato con la presidenza del Consiglio regionale. Ora, a seguito dell'inchiesta "Farmabusiness", proprio sui lati oscuri della sanità calabra, è detenuto con questa accusa. Grazie all'operato dell'onorevole Tallini il gruppo criminale Grande Aracri ha potuto ottenere facilitazioni, contatti e incontri con funzionari della Regione per ottenere agevolazioni. Per questo motivo gli viene contestato il concorso esterno e viene considerato la cerniera tra i clan e la pubblica amministrazione. Si può scegliere se si vuole andare oltre l'occasione di speculare e armare una polemica che per la gran parte è strumentale e con questa bloccare...

intervengo molto rapidamente perché credo che questa discussione vada fatta in un modo e in un contesto diverso, ricostruendo un quadro. In questi mesi abbiamo avuto sollecitazioni da molti (Forze dell'ordine, magistratura, commercianti, realtà imprenditoriali) che ci hanno spiegato quanto la lotta alla mafia in questo momento assuma un valore ancora più particolare di prima, perché il rischio reale che le mafie possano approfittare della crisi economica che la pandemia ha prodotto è molto grave e molto rilevante. Consentitemi di dire che se la risposta della politica e del Parlamento è questa discussione, penso che sia totalmente inadeguata

che i toni e il contenuto di alcune dichiarazioni del presidente Morra erano sbagliate e che le parole erano adatte a chi rappresenta un'istituzione. Detto questo, Presidente, se la situazione è quella di cui ho discusso, penso che dobbiamo cambiare registro la discussione non si possa esaurire in una polemica o in un braccio di ferro ma debba guardare alla priorità di noi tutti, ossia combattere le mafie e che - lo dico a tutti, non do la responsabilità a qualcuno - delegittimare, svuotare e boicottare la Commissione antimafia, facendo venir meno uno strumento decisivo

offeso da alcune dichiarazioni che nulla hanno a che fare con la lotta alla mafia e che hanno offeso la memoria di Jole Santelli) e tutti noi a guardare a questa priorità,

cerchiamo di aprire una discussione e vediamo su cosa è possibile ragionare per rilanciare il lavoro della Commissione antimafia (lo deve fare prima di tutto il Presidente). Invito tutti a fare un passo indietro; mettiamoci a disposizione di una priorità che abbiamo come politici di destra e di sinistra, al Governo o all'opposizione: combattere le mafie e mettere nel mirino la criminalità organizzata. *(Applausi)*. Le nostre polemiche non devono andare a condizionare negativamente la lotta alla mafia. Davvero

Moro utilizzava sempre un'espressione: «La persona prima di tutto». che proporre che il Presidente della Commissione antimafia

mandando al Paese un messaggio chiarissimo: ovvero che la persona non vale per quello che è ma per quello che ha o che può dare. E questo è inaccettabile perché nessuno di noi sa né il momento, né l'ora, né il modo. Quindi, il fatto che Jole Santelli fosse purtroppo malata di cancro, o che potesse essere un'anziana o una persona con disabilità, avrebbe determinato l'impossibilità di una sua candidatura? in questo caso come in altri, nelle decisioni legislative e proposte emendative a volte è sottesa questa sottile visione della nostra società.

sarebbe opportuna quantomeno una parola di profondo rammarico per un'espressione volgare, usata come metafora politica, quella relativa alla riverginazione dell'imene.

come Morra avrebbe potuto utilizzare. Poi ho ascoltato l'intervento del senatore Endrizzi. È vero: le accuse in capo al presidente del Consiglio regionale della Calabria Tallini sono molto gravi e bisogna considerarle nella gravità dell'accusa (che è un'accusa) e nella gravità del contesto. Però quell'intervento perde un orientamento politico laddove il MoVimento 5 Stelle e il Governo hanno riconfermato a capo dell'ENI non un indagato ma un imputato (stando alla procura della Repubblica e alle sue accuse) per la più grande tangente internazionale mai pagata dall'ENI. Quella non è un'indagine: lui è un imputato e a breve si dovrebbe arrivare a sentenza. Forse per prudenza io non l'avrei riconfermato, perché potrebbe accadere quello che è accaduto per l'amministratore delegato della Leonardo SpA, ex Finmeccanica, condannato

credo che anche in quest'Aula ci siano diversi malati oncologici, anche a distanza di pochissimi metri dal sottoscritto. E credo che chi mi conosce (e non solo) capisca che tutti quanti noi italiani, tutti, proprio perché ognuno potrebbe aver sperimentato su di sé l'esperienza amara del dolore vissuto da chi ti sta accanto, portiamo rispetto nei confronti di chi combatte la malattia, qualunque essa sia. Esiste una questione che si chiama rispetto. Io ho ascoltato tutti. Ricordo a me stesso che la defunta Jole Santelli, in un'intervista rilasciata ad un quotidiano cosentino

Vi invito a verificare. Ora, io devo chiedere scusa a tutte quelle persone che, avendo sperimentato sulla loro carne la sofferenza di una malattia imponderabile, di una malattia lancinante, che non ti dà la possibilità di costruire futuro, hanno avvertito in quelle parole un'offesa alla loro condizione. A quelle persone io devo chiedere scusa, perché, comunque, avendo pronunciato una frase sincopata, cioè senza aver completato il pensiero, ho prestato il fianco a tutte le interpretazioni possibili.

Un poco, però, ci conosciamo, signor Presidente, e, se una cosa contraddistingue la mia azione politica, è quella di guardar sempre a chi sta dietro di me, a chi è più debole, più fragile, più sofferente. Io sono un senatore eletto in Calabria e mi vergogno per le condizioni in cui versa la sanità calabrese.

alcuni fatta sapientemente, con l'abilità del sarto: prendo qualcosa di qua, prendo qualcosa di là e poi costruisco qualcosa di assolutamente diverso rispetto all'originale

nonché un cittadino, nonché un congiunto di persone che hanno dovuto fare i conti con la sanità pubblica calabrese, dovendo scappare e dovendo anche andare fuori Regione perché, altrimenti, non c'erano problemi nel senso che tutto si risolveva male. Io stesso ho prodotto, nella passata legislatura ma anche in questa legislatura, interrogazioni parlamentari, alle quali non ho avuto risposta, per casi di malasanità, cui è seguita, probabilmente, anche malagiustizia, perché in Calabria si muore anche di questo. Se io allora allora ho di fronte un quesito, che recita: secondo lei, senatore Morra, la Calabria è irrecuperabile? E la mia risposta è: la Calabria è irrecuperabile nella misura in cui il Governo centrale decide di non investire in formazione, istruzione e cultura; perché questa è stata la mia risposta, io non sto affatto asserendo che la Calabria sia condannata ad un destino tragico, come parecchi vorrebbero. *(Applausi)*. Io sto semplicemente mandando un grido disperato di aiuto alle istituzioni, anche al mio Governo, perché lo supporto anche io, che ancora oggi ha difficoltà ad indicare un Commissario *ad acta* per la sanità calabrese. Vedete, adesso sto portando un argomento che potrebbe tirare la volata alle cosiddette opposizioni, perché io ho un solo padrone: si chiama verità. Ed è questa la verità, che parecchi non vogliono sentire. Allo stesso modo, signor Presidente, è altrettanto vero che c'è un'altra verità, cioè che in Calabria, se si indaga sui rapporti perversi fra sanità pubblica e sanità convenzionata, molto spesso si scopre l'indicibile, come appunto è stato dimostrato... "Farmabusiness"*,* condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro la volta passata. È altrettanto vero, signor Presidente, che io ho l'obbligo morale - di fronte al quale non mi sono sottratto - di chiedere scusa a tutte quelle persone che autenticamente e sinceramente

Chi è che ha delle responsabilità su quanto avvenuto? Ricordo poi a tutti che, durante la campagna elettorale per le ultime regionali, la stessa Jole Santelli, con un coraggio e con una determinazione che le vanno comunque riconosciuti, in più interviste, anche ad Antonello Caporale su «Il Fatto Quotidiano», ebbe a prendere in considerazione il tema della malattia, avendo il coraggio di portarlo al centro del dibattito pubblico, cosa che con grande ipocrisia e tanto perbenismo italico, ipocrita e dai sepolcri imbiancati, non è concesso. Se allora lei ben ricorda, Presidente, in occasione della commemorazione di Jole Santelli, fu il sottoscritto a intervenire in Aula, pregando tutte le forze politiche di lavorare*.

con lei la Calabria ha perso un riferimento e una guida, anche rispetto a quel concetto di legalità che oggi è stato più volte richiamato.

La relatrice, senatrice De Petris, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

arrivare qui non solo con un dibattito generico ma mettendo a disposizione di questa lotta uno strumento assolutamente fondamentale.

iniziative sempre più adeguate e necessarie a difendere le donne nella lotta contro la violenza e anche per avere tutti

Il disegno di legge in discussione, approvato all'unanimità dalla 1a Commissione, rappresenta un importante tassello nel quadro complessivo della lotta dello dello Stato contro la violenza di genere, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica. *(Brusio. Richiami

su un fenomeno gravissimo qual è quello della violenza di genere e del femminicidio, che purtroppo non sembra conoscere soste né arretramenti. La violenza basata sul genere è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Le Nazioni Unite, in occasione della Conferenza mondiale sulla violenza contro le donne, tenutasi a Vienna nel 1993, definiscono tale violenza come ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferenza della donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o l'arbitraria privazione della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata (articolo 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne). Secondo l'Istat, nel nostro Paese una donna su tre subìto una qualche forma di violenza nel corso della sua vita, specialmente in famiglia. Questo vuol dire che in Italia poco meno di 7 milioni di donne tra i sedici e i settant'anni hanno subito violenza fisica, dalle forme meno gravi a quelle più più gravi, come il tentativo di strangolamento o lo stupro. La punta dell'*iceberg* del fenomeno - lo sappiamo bene - è il femminicidio, che rappresenta una parte preponderante degli omicidi di donne, con la caratteristica della maturazione in ambito familiare o all'interno delle relazioni sentimentali meno stabili. L'Organizzazione mondiale della sanità ha reso noto da tempo che la prima causa di uccisione nel mondo delle donne tra i sedici e i quarantaquattro anni avviene per mano di persone conosciute. I numeri sono spaventosi: circa 140 casi all'anno in Italia per un totale di circa 600 femminicidi ogni quattro anni. Dal 2000 a oggi le donne uccise in Italia sono state più di 3.300, di cui 2.400 in ambito familiare e circa 1.650 per mano del proprio coniuge, *partner* o ex *partner*. Ciò significa che nel nostro Paese in media ogni tre giorni circa viene uccisa una donna. Nel 55,8 per cento dei casi tra autore e vittima esiste una relazione sentimentale, in atto al momento dell'omicidio o pregressa. Se a questi si aggiungono i casi in cui tra autore e vittima esisteva una relazione di parentela, si scopre che in più del 75 per cento dei casi le donne muoiono nell'ambito familiare di questa stretta cerchia, all'interno cioè dell'ambiente nel quale dovresti sentirti più sicura e più amata. All'interno della classe di femminicidi avvenuti per mano del *partner*, dei casi evidenzia che la vittima e l'autore sono coniugi o conviventi, il 12 per cento fidanzati, il 24 per cento aveva comunque intrattenuto una relazione sentimentale. Come era prevedibile, durante il *lockdown* della scorsa primavera la situazione si è ulteriormente aggravata: il numero complessivo degli omicidi è diminuito, ma non gli assassinii con vittime di sesso femminile. È questo uno dei dati più significativi che emerge dal *report* elaborato dal Servizio analisi criminale della direzione della Criminalpol. Il documento analizza infatti l'andamento dei reati riconducibili alla violenza di genere nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2020, confrontato con l'analogo periodo dell'anno precedente. Un approfondimento riguarda proprio i dati sugli omicidi volontari, che si confermano in calo rispetto a quelli dell'anno scorso; ma le vittime di sesso femminile aumentano, da 56 a 59

ne sono state vittime 44 donne e 14 uomini. Ciò significa che durante il *lockdown* ogni due giorni una donna è stata uccisa in famiglia. La violenza di genere, pur essendo, come abbiamo visto, un fenomeno strutturale e diffuso, resta però in gran parte sommersa. I dati che ricordavo prima, così impietosi, impongono allo Stato di dotarsi di strumenti per comprendere quali siano i meccanismi che legittimano e alimentano la violenza sulle donne e di elaborare strategie e politiche per contrastarli. In Italia la mancanza di dati statistici ufficiali aggiornati sul numero dei delitti commessi a danno di donne e, più in generale, sul fenomeno della violenza di genere è stata più volte posta alla nostra attenzione. La direttrice generale dell'Istat, Linda Laura Sabbadini, parlando nel 2019, durante la sua audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, ha proprio evidenziato come gli strumenti di analisi siano attualmente insufficienti e le fonti esistenti siano plurime, frammentarie, carenti e perfino non definite univocamente. Anche le fonti di tipo amministrativo in ambito sanitario, giuridico e sociale non risultano ancora adeguate. oggi al nostro esame si propone di colmare le lacune presenti nel nostro ordinamento, partendo da quanto disposto in merito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che definisce chiaramente le strategie che gli Stati aderenti devono porsi, con l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere. Le riassume nelle cosiddette tre P: prevenire, proteggere e perseguire, cui si aggiunge una quarta P P relativa alle politiche, asse strategico trasversale per la costruzione di un sistema integrato di raccolta di dati e di attività di monitoraggio e valutazione. In quest'ottica la Convenzione di Istanbul ritiene fondamentale che ogni Stato aderente si doti di strumenti in grado di effettuare una compiuta analisi dei complessi fenomeni sociali che stanno a monte dello scatenarsi della violenza e, infatti, all'articolo 11,

pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione». Quindi, noi con questo disegno di legge attuiamo esattamente ciò che la Convenzione di Istanbul aveva prescritto. Nell'articolo 1 si individuano le finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne. L'articolo 2 prevede che, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvalga dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istat L'Istat e il Sistan realizzano, quindi, con cadenza triennale un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca anche - questo è molto importante - stime sulla parte La disposizione assegna al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione dell'esigenza di rilevazione statistica

sulla violenza psicologica ed economica per le donne, che devono essere integrati anche con domande relative alla presenza dei figli minori. È previsto, inoltre...

sulla sicurezza delle donne effettuate dall'Istat, con la possibilità che gli stessi possano essere integrati dall'Istat e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, con appositi provvedimenti. Con l'articolo 3 si stabilisce che la relazione al Parlamento sull'attività dell'Istat, di cui all'articolo 24, venga integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2. Molto puntuali sono poi gli obblighi previsti

entro dodici mesi dall'approvazione di questo disegno di legge, metta in campo un decreto per far sì che il centro di elaborazione

per l'esecuzione del codice di procedura penale in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato. L'articolo 7 realizza indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati

Signor Presidente, solo poche parole per riconoscere l'importanza di aver portato proprio oggi in approvazione un disegno di legge che va a colmare la carenza delle strategie che, come Paese, possiamo mettere in campo. Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne arrivare oggi ad assumere un impegno così importante significa certificare che le istituzioni del nostro Paese non solo celebrano questa giornata nel doveroso ricordo e nella testimonianza delle vittime di violenza, ma si assumono la responsabilità fattiva di mettere in campo politiche che vadano a contrastare questa violenza senza se e senza ma. Il processo di conoscenza di cui ci andiamo a dotare grazie a questo provvedimento, non riconosce alla

per aver portato questo provvedimento in Aula, sono grata alla relatrice per averlo seguito con così grande attenzione in Commissione e a tutte le forze politiche che, in modo trasversale, l'hanno sostenuto. Le politiche che metteremo in campo a partire da questo provvedimento si dovranno rivolgere certamente alla prevenzione, alla protezione, al perseguimento dei reati ma, ancora e sempre di più, a promuovere quella libertà e quella dignità che dobbiamo restituire a tutte le donne del nostro Paese e che solo una piena parità di genere potrà realmente tutelare e garantire. Sia oggi questo un punto di partenza ulteriore per un percorso da fare tutti insieme come istituzioni e come Paese.

in sede redigente alla 2ª Commissione permanente

È molto importante che il Senato la celebri con l'approvazione da parte dell'Assemblea del disegno di legge recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. Ringrazio la Commissione tutta, la sua Presidente e in particolare...

di cui all'allegato A del disegno di legge, rispetto a tutti i reati elencati al comma 3 dell'articolo 5, poiché è mia opinione che questo Parlamento, con il presente disegno di legge, possa fare la differenza, ovvero segnare un punto importante verso una maggiore emersione del fenomeno. È stata più volte citata la Convenzione di Istanbul, che fa riferimento alle tre P (prevenire, proteggere, perseguire) per addivenire a una quarta P, quella relativa alle politiche. Per prevenire bisogna anche proteggere, e mi rifaccio ai centri antiviolenza, ottima intuizione della politica, sperando che non restino senza fondi adeguati. dicevo, proprio con particolare attenzione alla relazione vittima-autore, svolgono un ruolo insostituibile i centri antiviolenza, che da sempre si pongono l'obiettivo di accogliere, ascoltare, protegge e, non da ultimo, orientare le donne vittime di violenza. È sui centri antiviolenza che le istituzioni devono puntare, fornendo tutto il supporto necessario poiché rappresentano lo strumento senza il quale molte donne non riuscirebbero neanche a trovare il coraggio per rompere le catene che le legano ai propri carnefici. È all'interno di tali centri che donne abusate psicologicamente prendono coscienza di ciò che hanno vissuto, perché non dimentichiamoci che quando si subiscono cooptazioni psicologiche si rinuncia persino al proprio punto di vista pur di sopravvivere e si arriva a pensare che ciò che si subisce è normale. È proprio attraverso percorsi mirati ad incrementare l'amor proprio e l'autostima che queste donne realizzano il male subito e smettono di compiacere, finanche giustificandolo, il proprio carnefice. Non bisogna fermarsi, ma perseguire nell'intento di creare tutte le occasioni necessarie per combattere il fenomeno. La politica è presente ed anche il disegno di legge di oggi lo dimostra, ma per creare le condizioni e per cercare di limitare il fenomeno tutti devono fare la propria parte. Quest'anno è senz'altro una ricorrenza che assume un significato ancora più forte: siamo infatti nell'era della pandemia da coronavirus e questa ha impattato pesantemente sul fenomeno della violenza domestica sulle donne e sulle ragazze, che sta letteralmente esplodendo proprio in ragione del *lockdown*. Nell'anno della pandemia incredibilmente diminuiscono gli omicidi, ma i femminicidi continuano la loro impennata, triplicati nei giorni del *lockdown*. I numeri ufficiali della polizia criminale raccontano che il 75 per cento delle vittime dei delitti compiuti in famiglia è composto da ragazze, mogli ed ex fidanzate. La pandemia ha abolito la socialità, ma non certo la violenza sulle donne: l'ha solo confinata ancor più dentro Siamo davanti ad un'emergenza nell'emergenza che cresce all'interno delle nostre abitazioni, è vero, ma che corre anche e soprattutto sul *web*. Proprio quel *web* deve essere la prossima imminente mira di questo Parlamento. C'è un forte bisogno di renderlo sicuro e controllato; a noi il compito di essere responsabilmente gli strumenti normativi a È proprio da quella rete che sovente oggi escono i mostri che entrano dentro le case delle donne, delle ragazze e non solo; è cosa nota infatti che reati come lo *stalking*, ad esempio, trovino il loro *incipit* proprio sul *web*, così come attraverso il *web* si consumano reati come il *revenge porn*, una tra le più vigliacche forme di violenza, che statisticamente vede come vittime principali le donne. Esso può ritenersi purtroppo un fenomeno in crescita esponenziale negli ultimi anni nel nostro Paese, dove gli episodi di vendetta pornografica e i ricatti sessuali hanno talvolta assunto contorni

dal dolore; proprio così, perché siamo nel campo delle cosiddette violenze invisibili, ferite che non perdono sangue, perché l'anima è l'unica ad essere colpita. Attraverso quel *web* il distacco emotivo del carnefice rispetto alla vittima è massimo, come se attraverso quello schermo passassero le immagini, passassero le parole digitali, ma mai le emozioni. Quel *web* oggi deve essere attenzionato dal Parlamento, con la stessa premura che si sta ponendo all'odierno disegno di legge, perché futuri interventi normativi divengano corollario e completamento di questo provvedimento, gli utenti della rete e responsabilizzando i genitori, perché competenza digitale ed educazione digitale non sono in alcun modo l'una sinonimo dell'altra e devono far parte entrambe del bagaglio culturale di noi tutti, adulti e ragazzi, nessuno escluso. Del resto lo stereotipo vuole che il *web* *web* inteso come un oggetto sia fortemente superato: il *web* è un luogo a tutti gli effetti, è luogo sconfinato e senza protezione. Io da donna ad essere sincera quella assenza di protezioni in rete l'avverto in maniera nitida. L'insulto, l'*hate speech* e la minaccia sono dietro l'angolo, pronti ad essere lanciati contro un popolo di odiatori e di mazzieri del *web* e se sei donna si perde anche il limite. Le donne abusate e violentate assomigliano a fiori recisi - questa è l'immagine che mi sovviene - e come fiori recisi sono destinati ad appassire prima. È la loro anima che appassisce, prima ancora che il corpo. È il dolore che le attraversa a spegnerle e ogni donna che si spegne rappresenta un fallimento per le istituzioni e per la società tutta. Mi sento di dire che questo Parlamento non fallirà, non perderà l'occasione per fare la sua parte nella storia

colleghe e colleghi, il mio percorso politico è iniziato nel 1999, quando sono stata eletta presidente del Comitato per le pari opportunità del Sud Tirolo. All'epoca eravamo molto attive nella battaglia per i diritti delle donne e abbiamo fatto molte campagne per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

All'epoca queste campagne suscitarono grandi discussioni e molti uomini si dissero offesi da tali rappresentazioni. A vent'anni di distanza ho l'onore di parlare di questi temi in Senato e mi sembra che nulla sia cambiato. Oggi quelle campagne, probabilmente, non susciterebbero più scandalo e tutte le più alte cariche dello Stato si esprimono pubblicamente contro la violenza sulle donne, ma il fenomeno non si è arrestato e, anzi, i numeri ci dicono che la situazione è peggiorata, con 93 femminicidi solo quest'anno, di cui due proprio in queste ore. ore. Ci si chiede allora come tutto questo sia possibile, nonostante le campagne, l'attivismo delle femministe e le leggi, che nei vari Paesi europei hanno inasprito le pene. L'unica risposta è che il maschilismo è un principio fondativo delle nostre società e ha radici talmente profonde, che ci vorranno davvero tanto tempo e tanti sforzi prima di rimuoverlo della nostra cultura. È chiaro che se l'uomo, nel suo inconscio, crede di essere superiore alla donna e questa poi si ribella, non facendo quello che vuole lui, o addirittura aspira a una vita senza di lui, spesso egli reagisce nell'unico modo che ha disposizione, ovvero la violenza. Quindi, ciò che principalmente c'è da fare è contrastare questa cultura di presunta supremazia maschile, che troppo spesso trova alimento nei *mass media*, dalla pubblicità alla rappresentazione della donna nelle serie televisive.

che chiama la maestra per spingerla a lasciare il lavoro; tutti discutono di cosa fa questa donna nel suo privato e nessuno parla di chi ha commesso reati, dalla preside che l'ha indotta al licenziamento a tutti coloro che hanno condiviso i video. Per non dire poi della Rai: solo grazie alla protesta delle donne non è stata mandata in onda l'intervista all'uomo che ha sfregiato Lucia Annibali, spruzzandole dell'acido sul volto. Come ha ricordato Michela Murgia, a nessun ladro viene fatta un'intervista per sapere perché ha rapinato una banca. D'altro canto, a nessuno verrebbe mai in mente di pensare che la banca possa avere una qualche responsabilità per il furto che ha subito. Invece nelle donne, nelle vittime, l'opinione pubblica cerca sempre una colpa, come si può leggere nel commento di Vittorio Feltri sulla vicenda della diciottenne, che, mentre partecipava a una festa, è stata portata in una stanza, rinchiusa e violentata per una notte intera. Per Feltri la ragazza si è comportata da ingenua e per questo dice di voler concedere le attenuanti generiche alla vittima. Se non fosse stata ingenua, secondo la logica di Feltri, sarebbe stata pienamente colpevole. Questa cultura del «com'era vestita», del «perché è entrata nella sua camera da letto» e del «cos'ha fatto per far perdere la testa a uno per bene» è tanto radicata nelle menti delle persone. di noi donne, di noi femministe, quindi è proprio quello di rilevare i meccanismi invisibili della denigrazione delle donne, che si nascondono ovunque, anche nel linguaggio, che conosce la forma femminile solo per le posizioni basse, mentre quelle di spicco esistono solo al maschile, o in cui vengono usate metafore come quella della riverginazione dell'imene. Ecco l'aspetto più difficile della battaglia a questo insidioso fenomeno, ma naturalmente non è l'unico. Ci sono ancora lacune legislative che vanno colmate con urgenza: il codice rosso ha introdotto nuove fattispecie di reato molto importanti come il *revenge porn*, ma il reato di istigazione all'odio di genere non ha ancora visto la luce. Tuttavia, la più grande cassa di risonanza della cultura maschilista e misogina è la Rete. Qui, in un clima di vera e propria impunità, l'odio contro le donne che non si comportano come qualcuno vorrebbe raggiunge i massimi livelli. Manca altresì una norma efficace contro la violenza economica. Sappiamo che quest'ultima è il terreno fertile per ogni tipo di violenza. In Italia l'occupazione femminile è la più bassa d'Europa e c'è un alto numero di casalinghe senza alcun tipo di tutela economica. In Austria e in Germania hanno diritto a una percentuale del reddito del marito, che possono ottenere con esecuzione forzata anche in costanza di matrimonio. Ci sarebbero tanti altri esempi sulle lacune del diritto di famiglia a danno delle donne, ma purtroppo la discussione da noi è solo intorno ai padri separati. Bene allora il provvedimento in esame che, col miglioramento delle statistiche, contribuisce a inquadrare meglio il fenomeno e può essere anche uno strumento importante per le decisioni della politica, politica, che deve lavorare per la parità, perché la lotta per la parità e quella contro la violenza sono due facce della stessa medaglia; deve favorire la presenza delle donne nei ruoli apicali e incentivare i padri a farsi carico del lavoro familiare. Alle donne la metà del mondo, agli uomini la metà della famiglia: questo dev'essere il nostro *Leitmotiv.* Ciò può essere raggiunto favorendo l'occupazione femminile, aumentando le strutture di accudimento dei figli, premiando i congedi parentali presi dai padri e prevedendo quote di genere nella politica e nelle posizioni di vertice della pubblica amministrazione e delle imprese quotate in Borsa. La politica e soprattutto le donne in politica sono chiamate ancora a un grande impegno per sconfiggere la pandemia delle tante forme di violenza contro le donne. Sarà un cammino lungo, ma solo alla fine l'Italia potrà davvero definirsi un Paese civile e moderno Signor Presidente, signor ministro Bonetti, sottosegretario Castaldi, oggi è il 25 novembre 2020 e purtroppo siamo ancora in quest'Aula a ricordare le donne che non ci sono più, che sono state uccise, e quelle che ci sono ancora, ma soffrono, perché sono state gravemente maltrattate.

il mondo almeno una donna su tre nel corso della propria vita subisce gravi forme di violenza e di mutilazione, fino a essere uccisa.

istituita sulla base dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, che dice di basarsi sui valori della non discriminazione e della parità tra uomini e donne. L'Italia, uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea,

è omogenea su tutto il territorio nazionale, trasversale e indipendente dal lavoro, dalla formazione e dal tipo di vita che le persone conducono; prescinde da tutto questo si basa su una discriminazione nei rapporti tra uomini e donne. Questo è confermato dai dati che già oggi l'Istat ci offre, perché l'80 per cento delle donne non subisce violenza dagli estranei, come magari i luoghi comuni vogliono farci credere, ma dai propri familiari,

ogni due giorni e mezzo. Quest'anno, durante il *lockdown,* quando le donne sono state segregate in casa insieme agli uomini autori di violenza, abbiamo registrato un femminicidio ogni due giorni, quindi con una frequenza

La Convenzione di Istanbul è una pietra miliare sotto moltissimi profili. Nel 2011 è stata votata dal Consiglio d'Europa e ratificata in Italia nel 2013.

indica la strada per contrastare la violenza di genere. Ci dà quattro linee guida strategiche e ci dice che bisogna attuare leggi sulla prevenzione, sulla protezione, sulla punizione e sulle politiche, cosa che stiamo facendo. Oggi lavoriamo sulla quarta P, ossia sulle politiche. Sulla prevenzione lavoreremo con altri disegni di legge che la Commissione sul femminicidio e le colleghe stanno preparando, perché bisogna lavorare nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa l'università, che forma i giudici, gli avvocati, i giornalisti (così da non leggere più cose come quelle che abbiamo letto ieri su «Libero»), «Libero»), la classe dirigente che deve cambiare la cultura di questo nostro Paese, i pubblicitari, coloro che passano le immagini e coloro che devono formare una nuova coscienza critica in questo Paese. Quanto alla protezione, storiche sono le battaglie e l'importanza dei centri antiviolenza, mentre meno storico, ma molto efficace, è il ruolo dei centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti. Dobbiamo dire chiaramente

In tema di punizione è stato fatto molto. Molti riconoscono che l'Italia ha un sistema giuridico completo. Anche con l'ultimo codice rosso sono stati integrati i reati che la Convenzione di Istanbul prevedeva, come il *revenge porn*, il reato di deturpazione del viso, il matrimonio coatto e le mutilazioni genitali femminili. Abbiamo un sistema giuridico completo,

a partire dai pronto soccorso, dalle Forze dell'ordine, dalle questure, dalla magistratura, dai centri antiviolenza e dai centri per gli uomini maltrattanti, devono confluire in un'unica grandissima banca dati che arriva all'Istat, la quali li rielabora e li consegna alla politica, affinché possa attuare le politiche migliori, più efficaci e mirate per contrastare questo fenomeno. Abbiamo bisogno di

Possiamo fare tutto questo solo se ci diamo lo spazio, nel tempo, per non dire ogni volta che arriviamo in Aula: ancora un disegno di legge sulle donne; certo, ancora; fino a che non avremo attuato la Convenzione di Istanbul in tutte le sue quattro linee guida, non avremo finito di fare il nostro lavoro né di completare tutta l'azione strategica che ci serve per debellare la violenza in Italia. *(Applausi)*. Siamo pronti a lavorare duramente, giorno per giorno; è quello che stiamo facendo in Commissione femminicidio, con la guida, l'aiuto, la collaborazione e la grande unità di intenti del ministro Bonetti.

a farlo gli uomini, certamente quelli maltrattanti, ma anche i non maltrattanti e i non violenti, che devono aiutare quelli violenti a cambiare radicalmente le loro parole, il loro comportamento e il loro modo di stare nella società che vogliamo costruire.

merita, chiede e pretende. Anche quest'anno, derogando alle regole che ci siamo dati, abbiamo giustamente inserito il disegno di legge in discussione in coincidenza con questa giornata. Questo disegno di legge è il figlio

devo dire anche con qualche fatica e, a volte, qualche contrapposizione, superando talvolta le differenze di visione tra noi. Non casualmente compaio come seconda firmataria, dopo la collega Valente

dalle prime riunioni della Commissione abbiamo sottolineato proprio ciò che il titolo di legge recita, ovvero «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere». Noi, cari colleghi, abbiamo aggredito così un nodo antico e annoso, ovvero l'assenza dei dati e di banche dati che potessero dialogare tra loro a livello nazionale, ma anche europeo. La raccolta dei dati non è una mania della matematica, ma l'esigenza di una dimensione quali-quantitativa per restituire analisi statistiche reali, utili ed efficaci. È questo il senso del nostro disegno di legge.

tra i quali la cadenza triennale delle ricerche di campionatura dell'Istat e la cadenza biennale delle indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio e ancora la relazione tra vittima e autore della violenza. Tutto questo perché? Abbiamo il dovere di far emergere un sommerso, quello della violenza. Sappiamo quanti di questi atti di violenza scivolino e si nascondano nelle lesioni, nelle percosse, nelle minacce

ragionati, a livello interministeriale, che riguardano anche i casi di denunce per violenza subita, ma anche di femminicidio, ovvero quegli omicidi di donne in ragione del loro essere essere donna. Insomma, l'obiettivo che ci siamo dati e che oggi in qualche modo raggiungiamo - o, comunque, il percorso che abbiamo - è un sistema informativo sulle violenze di genere, per mettere per mettere a punto politiche di prevenzione e di contrasto, proprio per non fermarci a quella punta dell'*iceberg* e far emergere lo spazio invisibile e maledetto delle violenze domestiche o che si annidano e si nascondono dietro le relazioni sentimentali private

giornata non per vuote celebrazioni, ma per ricordare tutte le vittime di violenza nel mondo e per richiamare l'attenzione

indossare questa mascherina, come campagna di sensibilizzazione, richiamando anche quello che è successo durante il *lockdown* e contestualizzandolo. Non sfuggirà a nessuno, che la situazione di pandemia che stiamo vivendo ci deve spingere a riflettere maggiormente sulla ricaduta sul mondo femminile, anche in termini di crisi economica, di tenuta, di coesione sociale e di condizione occupazionale. Mezzo milione di donne ha perso il lavoro in questi ultimi mesi e per questo pensiamo che proprio le famiglie, insieme alle donne, stiano pagando il prezzo esistenziale più alto alla pandemia. Occorre dunque un'attenzione politica e istituzionale di tutti, che non si esaurisca nelle celebrazioni di oggi, ma si concretizzi in un sistema organico di misure straordinarie e di tutela e in un piano di strumenti economici e ristori, nonché nell'applicazione integrale delle norme penali previste per rendere giustizia alle vittime e punire gli autori dei reati. quindi di una battaglia politica quotidiana, ma anche culturale, contro ogni arretramento che favorisce e fomenta tutte le forme di violenza sulle donne, senza se e senza ma, com'è stato detto; aggiungo: senza *copyright* politici da parte di nessuno. È una questione sociale che riguarda tutti, non un fatto privato, e non è appannaggio di nessuno. Per questo il nostro pensiero va oggi a

né lasciamo mai loro l'onere della prova della violenza subita. Purtroppo, diciamocelo, quello di cui stiamo parlando è un mondo che attraversa il mondo, le geografie, le latitudini, le religioni, i ceti e le credenze. È un flagello sociale e una pandemia nella pandemia, che, come tale va guardata e percepita, senza girarsi mai dall'altra parte. I dati ci dicono infatti che ognuno di noi conosce almeno un caso di violenza: se non lo vediamo, vuol dire che abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo girato le spalle, e questo ci rende complici. Dobbiamo tutti assumere la questione come un'emergenza sociale, collettiva e condivisa, non come un fatto privato da scaricare sulle spalle delle vittime.

diventa obbligatoria l'indagine nel rapporto tra autore e vittima. In ogni caso, questa è anche l'occasione per fare una riflessione di carattere generale. Non aggiungo nulla alle cose che ho già ascoltato e procedo rapidamente, anche in relazione alle esigenze

le mura di casa, che dovrebbero essere invece il perimetro della protezione di ciascun individuo, a maggior ragione di ogni donna di questa società. Dobbiamo prenderci un impegno: non deve accadere mai più

stato ricordato, qui mettiamo un mattoncino per rafforzare l'impegno che abbiamo assunto dentro la cornice della Convenzione di Istanbul.

facciamo la nostra parte per rafforzare quel quadro. Lo dico innanzitutto a lei, signor Ministro, che molto si è spesa in questa direzione: abbiamo fatto molto in questi anni, a partire ad esempio dal tema della punizione, ma molto dev'essere ancora fatto, soprattutto se penso a quel pezzo importante dell'ossatura dell'intera strutturazione che fa parte della strumentazione per contrastare la violenza di genere, ossia le case rifugio e i centri antiviolenza. Molto è stato fatto a questo proposito in termini di risorse, di risorse, anche in termini di aggiustamento rispetto a un meccanismo più intelligente di quello che si era immaginato in passato rispetto alla ripartizione dei fondi attraverso le Regioni. Molto dev'essere ancora fatto, però, perché non c'è dubbio che la loro entità, ma soprattutto la possibilità che possano essere finanziate con una prospettiva più lunga sul piano temporale, siano l'unica garanzia per programmare i lavori e le attività di quelli che sono diventati terminali importantissimi in questa battaglia per il contrasto alla violenza sulle donne. Questo è un impegno che ci siamo assunti, che abbiamo portato avanti e che bisogna

democratica di questo Paese venga scaricata innanzitutto sulle spalle delle donne e che siano esse innanzitutto a pagare il prezzo più alto. Lo dico perché non ci stiamo misurando con disuguaglianze nate oggi:

sperimentando fino in fondo, che però rischiano di essere una trappola insidiosa per molte donne in assenza di un quadro di regole, a partire, ad esempio, dal diritto alla disconnessione.

finestra"). Devo purtroppo annunciare che è scomparso Maradona, lo sportivo, il calciatore che

Signor Presidente, anch'io, come il senatore Laforgia, parto da ringraziamenti non formali. Non è un tempo facile per arrivare in Aula con un provvedimento votato all'unanimità e il dibattito di questo ne è una prova; però ci siamo riusciti e, se l'abbiamo fatto, ovviamente è merito di tutti (di nessuno in particolare, ma di tutti in egual misura). Parto ovviamente dai ringraziamenti ai rappresentanti del Governo:

quelli competenti. Mi consentirete poi un ringraziamento particolare a tutti i componenti e le componenti della Commissione che ho l'onore di presiedere: a tutti, maggioranza e opposizione. Come sottolineava la senatrice Rauti, Rauti, insieme ai due vicepresidenti, ieri abbiamo tenuto un'importante iniziativa e abbiamo davvero lavorato tutte insieme. Questo credo sia un merito soprattutto da ascrivere al tema di cui siamo chiamate ad occuparci. Un ringraziamento particolare rivolgo anche ai componenti e alle componenti della Commissione affari costituzionali e al presidente Parrini e uno speciale, da donna a donna, a una relatrice combattente, com'è sempre la senatrice De Petris, che non si è mai arresa di fronte alle tante difficoltà che abbiamo incontrato. Credo che gran parte del merito di essere arrivati oggi in Aula sia suo, più che di tutti noi, quindi grazie davvero.

70 femminicidi o 90 non sono la stessa cosa; in mezzo ci sono 20 persone, 20 famiglie, 20 donne, 20 storie dolorose e drammatiche. Non mi sentirete dare i numeri, quindi. Non li darò perché questo Paese non ne dispone e per questa ragione abbiamo pensato di approntare questo disegno di legge, che chiede innanzitutto di fare sui numeri, monitoraggi costanti per osservare il fenomeno nel corso del tempo, ma soprattutto di indagare il sommerso. Tanti tipi di violenza come quella psicologica ed economica non arrivano a galla. Lo facciamo chiedendo a tutti gli operatori di indagare quella famosa relazione tra autore e vittima

anche in altre circostanze in queste ore - con parole di verità, che credo debbano interrogare la politica, le forze politiche, ma soprattutto il Parlamento e il Governo di fronte a un dato che viene letto ed è semplice, che interroga e inchioda ciascuno di noi e la politica, in modo particolare, alle sue gravissime responsabilità. Noi abbiamo un quadro normativo oggi assolutamente soddisfacente. Lo posso dire assumendomi la responsabilità di quanto dico e non abbiamo nulla da invidiare ad altri Paesi europei. Siamo a ricordare a tutti noi

dal codice antimafia come il divieto di soggiorno in un Comune o l'obbligo di residenza in altro Comune, per tentare di aggredire il fenomeno. Abbiamo davvero dotato l'impianto normativo di misure dure.

perché, se non ci interroghiamo, non renderemo giustizia a noi stessi, alla nostra onestà intellettuale e, soprattutto, alle donne vittime di violenza e alle tante che ogni giorno lavorano su questo fronte. La cosa che non va

come una donna avrebbe potuto chiedere di più e meglio aiuto e sul perché non lo abbia fatto. Perché continuiamo a farci domande su cosa avrebbero dovuto fare le donne? Vorrei che provassimo a chiederci cosa può scattare nella mente di un uomo che si attribuisce il diritto di poter abusare di una donna senza che questa gli dia esplicitamente il proprio consenso. (*Applausi*). Quanto ha detto ieri Feltri non è una cosa che offende Feltri o una testata giornalistica. Deve essere un qualcosa che faccia interrogare noi tutti sul perché in Italia non ci sia stata una reazione corale di indignazione rispetto al fatto che una donna possa scegliere di andare vestita succinta a qualsiasi ora, possa uscire di casa a qualsiasi ora, possa andare a un festino dove si fa uso di coca o pensare di fare la *escort.* È una sua scelta, che sarà giudicabile se costituisce reato su altri fronti.

Il tema è la prospettiva. Proviamo a chiederci cosa scatta nella mente di questi uomini. Esiste ancora l'impalcatura di un modello patriarcale, che pensiamo di avere cancellato dalla carta e che per questo è più subdolo e pericoloso. Nei fatti quel modello è ancora fortemente vivo.

oppure devono fare tripli o quadrupli salti mortali facendo i conti con i loro sensi di colpa e con la difficoltà di condividere e conciliare la responsabilità familiare con quella pubblica. E lo fanno con grandissima difficoltà.

25 novembre dell'anno scorso ci ha detto esattamente questo: più della metà degli italiani pensa che una donna si è trovata a subire una violenza perché se l'è cercata o perché non l'ha evitata. È grave, gravissimo, ed è questo che ci deve indignare

Chiedo a tutti voi: quindi? Lei lo ha tradito: e quindi? Questo giustifica che un uomo ammazzi una donna? Perché lei lo ha tradito? Credo proprio di no. Giustificare in qualche modo o trovare delle attenuanti generiche in questo è un errore, è frutto di un pregiudizio e di uno stereotipo

storia, un sesso si è autoproclamato più forte dell'altro e ha deciso che a lui spettavano i compiti della vita pubblica e alle donne spettava essere angeli del focolare. Ci sono stati tornanti storici, civiltà questo non accadeva, quindi non è vero che c'è un sesso più forte e uno più debole. Io credo che le donne anche in questo frangente storico, nel corso della pandemia, abbiano dimostrato la loro straordinaria forza. E allora il tema è provare a riconoscere questa forza, nelle scuole, in famiglia, nelle agenzie educative e nelle università che formano i formatori, nelle quali si scrivono i libri di testo che sono ancora pieni di stereotipi. Lavoriamo per una società che sia in grado di superare stereotipi e pregiudizi e, soprattutto, in grado di riaffermare parità effettiva tra gli uomini e le donne, una società che faccia del rispetto dell'altro, dell'altro sesso, un fondamento non solo della nostra Carta costituzionale ma a tutti gli effetti perché tra quella parità formale citata dalla Carta e quella sostanziale che sostanziale che si concretizza ogni giorno nella nostra vita quotidiana, purtroppo, il passo è ancora troppo lungo e il prezzo finiscono per pagarlo le tante donne che subiscono violenza.

Ringrazio il Presidente della nostra Commissione di inchiesta e tutti i suoi componenti per aver sottoscritto la proposta di legge in materia di statistiche in tema di violenza di genere all'unanimità. Ad oggi, i dati non rappresentano adeguatamente la violenza di genere contro le donne, sebbene *stalking*, violenza sessuale e maltrattamenti possano certamente essere considerati reati spia. Ecco il principale obiettivo del disegno di legge che voteremo convintamente. Abbiamo sempre lamentato la carenza di sistemi informativi che potessero parlare tra loro, anche per tutelare i figli delle vittime. Questo disegno di legge impone al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi, tra le altre, informazioni sulla relazione tra vittima e autore del reato per misurare adeguatamente questo tipo di violenza: un passo avanti per una maggior tutela delle donne e dei loro figli. Altri passi dobbiamo fare per adeguare le politiche di prevenzione e contrasto a questi drammatici episodi. Approfitto della presenza del ministro Bonetti, che ha sempre partecipato e sostenuto le attività della Commissione e che ringrazio, per sollecitare altri temi che la Commissione ha molto a cuore. Mi riferisco, ad esempio, all'implementazione delle risorse per l'intero sistema di prevenzione e semplificazione, all'erogazione ai centri e alle case rifugio. La proposta di revisione in sede Stato-Regioni è di ripensare ai sistemi di trasferimenti plurimi delle risorse destinate ai centri e alle case rifugio per le tempistiche dell'erogazione dei fondi molto lente.

Dalla scorsa legislatura, anche nella relazione finale, mi sono impegnata per avere una mappatura nazionale dei centri e delle case rifugio; è stata presentata anche una relazione da parte della nostra Commissione di inchiesta. Ci vuole un'analisi della *governance* a livello territoriale dei sistemi di finanziamento, con particolare riguardo alla distribuzione delle risorse nazionali e regionali. Ci sono sempre ritardi nella distribuzione, ma da un rapporto del 2020 di ActionAid è risultato che, tre mesi da marzo a giugno del 2020 e di fronte a un 120 per cento in più di richieste di aiuto ai centri rispetto al 2019 per i ritardi di erogazione dei fondi molti centri non hanno potuto pagare gli stipendi alle operatrici per sostenere le spese di guanti, mascherine, senza possibilità di effettuare tamponi. Il ministro Lamorgese ha chiesto ai prefetti delle varie città una sorta cuscinetto di accoglienza; il Dipartimento per le pari opportunità ha promesso di accollarsi quelle spese straordinarie, ma oggi i fondi non sono arrivati e, con la seconda ondata di Covid e le varie chiusure,

stanziati per il 2019, e credo e spero che il Ministro a breve firmi il decreto per i 28 milioni previsti per il 2020. Un altro punto sta particolarmente a cuore, un punto legislativo, e cioè creare un protocollo di requisiti per l'accreditamento dei centri e delle case rifugio univoco su tutto il territorio nazionale, e controllare e monitorare il lavoro e i servizi che questi centri dovrebbero dare per la tutela delle donne e dei loro figli, perché abbiamo notizie di centri che non fanno quello per cui percepiscono i soldi. Ulteriore intervento legislativo, fondamentale sul procedimento, è la regolamentazione dell'affidamento dei figli. Sappiamo che i tribunali non si parlano, quindi spesso il tribunale dei minori dà l'affido congiunto a una coppia in cui la moglie ha chiesto la separazione e c'è una denuncia nei confronti del marito o del padre dei figli. Questo non va bene; lo chiediamo da anni. Dobbiamo implementare i punti più deboli del codice rosso, che è stata una grandissima conquista. Sono giusti i tre giorni come tempo della denuncia perché arrivi sul tavolo del pubblico ministero, ma non è giusta la lentezza del procedimento perché è il momento in cui la donna è più esposta alle violenze e alle ritorsioni. *(Applausi).* In conclusione, stiamo facendo molto, ma non abbastanza. Chiediamo un cambio di passo culturale, è vero,

È diventato abituale anche da parte di rappresentanti delle istituzioni usare un linguaggio crudo e violento - penso a molti *talk show,* a volte, purtroppo, anche in Aula che toglie dignità e che riceve consenso per la sua immediatezza, proiettando la propria rabbia contro un nemico che "se l'è cercata", esattamente come dicono di tante donne: se l'è cercata, per quello che pensa o che ha detto o che ha fatto; così dicono. Non basta essere contro la violenza; si deve essere coerenti nei propri comportamenti, soprattutto se si ha un ruolo pubblico. Si vuole e si deve insegnare nelle scuole l'educazione al rispetto. Ricordo ancora la "settimana rosa" istituita nel 2009 dal Governo Berlusconi, con i ministri Gelmini, Carfagna e Prestigiacomo, per insegnare ai bambini nelle scuole ad essere contro la violenza. Poi si è persa negli anni, forse perché non andava troppo bene o non so. Ebbene, se pretendiamo di formare gli educatori, di formare i professori e gli studenti universitari, non dobbiamo dare spettacoli mediaticamente indecorosi. È dalla comunicazione e dall'uso delle parole che si può cominciare a parlare di rispetto. È da ognuno di noi, dalla pratica quotidiana del rispetto e della dignità, che tutti possiamo cambiare le cose. *(Applausi)*.

rappresentanti del Governo, colleghi senatori, stamattina appena sveglia ho acceso la televisione e dopo pochissimi minuti è stata comunicata la notizia di due femminicidi: uno avvenuto in provincia di Padova e uno in provincia di Catanzaro; uno effettuato da uno straniero e uno da un italiano. Entrambi gli omicidi da *partner* ed entrambi in zona rossa. Questo deve obbligatoriamente imporci una riflessione, perché questo dimostra quanto purtroppo sia trasversale il problema. Durante il *lockdown* c'è stato un calo significativo delle denunce rispetto all'anno precedente, che però sono aumentate di colpo a maggio-giugno appena c'è stata data la possibilità di uscire di casa. perché al contrario degli omicidi, le cui vittime sono uomini e per i quali il rischio è rappresentato dallo spazio pubblico, per le donne il rischio di subire violenza è all'interno della famiglia. Da dati Istat del 2018 otto donne su dieci conoscevano il proprio assassino e in più della metà dei casi questo era il *partner* o l'ex *partner*. Solo cinque uomini (pari al 2,4 per cento) è stato ucciso da un *partner*, peraltro attuale, e nessuno da ex. Nel corso di questa legislatura molto è stato fatto per cercare di porre un argine a questa deriva omicida, con l'istituzione del numero antiviolenza 1522 e con l'approvazione del cosiddetto fortemente voluto dalla Lega, legge che obbliga la presa in carico e l'ascolto della vittima da parte del magistrato entro tre giorni dalla denuncia: un grande passo avanti dal momento che nel 63 per cento dei casi di femminicidio il carnefice è un recidivo, ovvero la vittima aveva già denunciato di essere stata molestata o maltrattata dallo stesso. stesso. Evidentemente non basta dal momento che sono ben 91 le vittime di femminicidio dall'inizio dell'anno: una ogni tre giorni. Con questo documento la Commissione di inchiesta sul femminicidio vuole strutturare un metodo, che solo il tempo ci potrà dire se adeguato o meno, per capire però quali sono le cause scatenanti di tanta cattiveria. La maturità e l'attenzione che questo Parlamento dà alla situazione violenta attuale si evince anche dalla mediazione che ha trovato in questo documento, dove tutte le forze politiche hanno dato il loro contributo anche nel sottolineare le criticità di talune domande poste nel questionario, domande le cui risposte potevano prestarsi a interpretazioni pregiudizievoli o fuorvianti. A tal proposito ringrazio le senatrici Valente, De Petris e la maggioranza tutta per aver accolto il nostro ordine del giorno volto a svolgere un'identica ricerca anche sulla violenza perpetrata ai danni degli uomini, il tutto a fine comparativo. Non è sicuramente una gara e nessuno ha mai sostenuto il contrario. Ricordo a noi tutti e in prima battuta a me stessa che le donne hanno un importantissimo ruolo nel futuro della nostra società che è l'educazione dei nostri figli, maschi o femmine che siano, che devono crescere imparando il rispetto per la persona: uomo, donna, grasso, magro, alto, basso, bianco, giallo o nero. insegnare loro che la propria libertà finisce quando invadono lo spazio di libertà altrui, far capire loro che le parole sono armi pericolose, qualche volta letali. Bisogna usarle sempre con attenzione. Purtroppo però non sempre questo accade e qualche volta lo scivolone vede protagonisti persone che dovrebbero essere esempio per la società. A tal proposito, ricordo a quest'Assemblea che più di un senatore ci ha lasciato per patologie tumorali durante questa legislatura e qualche collega che partecipa attualmente ai lavori sappiamo che ne è affetto e sta combattendo questa malattia. Bene, senza timore di alcuna smentita, affermo che il valore aggiunto prodotto da queste persone ai lavori del Senato è pari se non superiore a quanto prodotto da tanti altri e mi limito qui. *(Applausi)*. Noi mamme dobbiamo far capire ai nostri figli che la debolezza è umana e non si può sopperire con la violenza, sia essa fisica o verbale. Dobbiamo spiegare che piangere, per un maschio, non è un tabù e anzi, a volte, può essere un valore aggiunto. Dobbiamo far capire chiaramente che non basta essere dotati di pene e gonadi per essere uomo, ma lo si è quando si rispetta il prossimo. Concludo il mio intervento comunicando che l'approvazione del provvedimento in esame rappresenta il superamento effettivo del femminismo da salotto *radical chic* e il successo del pragmatismo. Per questo motivo,

La statistica, infatti, assurta alla dignità di scienza autonoma da appena un secolo, ha sempre offerto un valido supporto conoscitivo e programmatico per fenomeni complessi, come ha dimostrato già durante la prima guerra mondiale e poi nelle fasi successive del dopoguerra e proprio come sta facendo in questi giorni, per fronteggiare la crisi pandemica. La raccolta dei dati numerici, infatti, offrirà una base scientifica imprescindibile per qualsiasi intervento, permettendo una maggiore comprensione del fenomeno e un migliore funzionamento dei meccanismi di tutela per le donne, già operativi nel nostro Paese. L'ausilio della disciplina statistica migliorerà senz'altro la capacità di previsione e dunque di prevenzione del fenomeno violento, permettendo di agire d'anticipo. certo a questo momento conoscitivo dovranno affiancarsi un'accurata e capillare azione informativa, tramite le agenzie di comunicazione, che dovrà per forza di cose rinnovarsi nel linguaggio e nello stile comunicativo, come noto con piacere stanno già facendo importanti aziende, il cui *target* è il mondo dell'infanzia. di inchiesta ci siamo prefissati l'obiettivo di intensificare gli interventi educativi nelle scuole, già nei prossimi anni, con personale adeguatamente formato e con pianificazioni strutturali, posto il fatto che la violenza contro le donne è prima di tutto una questione culturale, che attraversa in modo trasversale tutti i ceti sociali e che affonda le proprie radici nel permanere dello squilibrio di potere e nella visione asimmetrica, esistente nei rapporti tra uomini e donne, spesso rinforzata dal permanere di una mentalità restia al cambiamento. Posto ciò, si è individuato nell'indagine statistica un formidabile strumento di contrasto e soprattutto di comprensione scientifica della realtà, permettendo, sulla base del dato numerico, anche l'emersione del fenomeno, che in buona parte sfugge, perché si consuma all'interno delle pareti domestiche. L'approccio al fenomeno non può restare legato a reazioni di tipo emotivo, ogni qualvolta la cronaca ci presenta un caso, suscitando rabbia o compassione, complice anche certa stampa, che insegue il sensazionalismo, ma che resta in superficie e che rischia sempre di scadere in una rivittimizzazione di chi già ha patito trattamenti degradanti o di chi addirittura ha perso la vita. È ora di passare all'attacco e di intervenire in anticipo, come dicevo prima, e il presente disegno di legge intende fare proprio questo: una raccolta sistematica dei dati numerici, a cui seguirà una lettura ragionata degli stessi e dunque la predisposizione di interventi fattivi. Dobbiamo essere tempestivi, giacché tra i tanti effetti negativi, conseguenti al *lockdown*, c'è pure l'acuirsi di tale fenomeno. Il disegno di legge persegue la creazione di un flusso informativo sulla violenza di genere adeguato per cadenza e contenuto, prescrivendo obblighi di rilevazione a tutti i soggetti pubblici, ma anche privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale inserita nel Programma statistico nazionale, che dispone altresì l'attuazione di tale rilevazione di oggetto nella relazione annuale al Parlamento, trasmessa dal Presidente del Consiglio, circa l'attività dell'Istituto nazionale di statistica. Si prevede poi che tale Istituto, insieme al Sistema statistico nazionale, vadano a realizzare con cadenza triennale un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza di genere contro le donne, con attenzione alla parte sommersa. Si prescrive altresì che tutte le strutture sanitarie pubbliche forniscano i dati e le notizie relative alla violenza contro le donne e che, per una serie di reati puntualmente numerati, sia tracciata una relazione autore-vittima, secondo una rilevazione alla quale concorrano sia il Ministero dell'interno che quello della giustizia; quest'ultimo è tenuto ad aggiornare conseguentemente la disciplina applicata dal registro delle notizie di reato. Ancora, il disegno di legge dispone che l'Istituto nazionale di statistica e il Sistema statistico nazionale assicurino la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditate. In particolare, ho ritenuto importante evidenziare nelle elaborazioni statistiche il dato relativo alle patologie psichiatriche di cui possa essere affetto l'autore del reato. dalla necessità e dal dovere di contrastare con efficacia le condotte dei maltrattanti e di apprestare una reale tutela alle vittime di tali reati. Un fenomeno che risulta sconosciuto è che sono scarsamente tutelate le stesse persone offese. offese. In presenza di patologie psichiatriche accade, infatti, che il soggetto non ne risulti affetto e rimanga a convivere all'interno del nucleo familiare, dando luogo alla violenza. Pertanto, una volta accertata la conseguente incapacità di intendere e di volere del maltrattante, al fine proprio di tutelare l'incolumità della persona offesa, viene richiesta un'urgente misura di sicurezza. Dunque, solo facendo emergere dati reali relativi a un fenomeno così allarmante si possono apprestare maggiori strumenti per garantire il recupero del maltrattante, proteggere le vittime e fare adeguata prevenzione. Concludo dicendo che il mondo maschile e quello femminile, così vicini ma allo stesso tempo così lontani, devono riprendere un dialogo costruttivo improntato sulla reciprocità, come avviene in moltissimi casi di coppie evolute. Questa reciprocità non può prescindere dalla conoscenza di esigenze e differenze fisiologiche innegabili tra i due sessi, ma che possono coesistere e armonizzarsi tra loro, senza nessuna sopraffazione. Il rapporto tra uomini e donne deve creare vita, non deve essere mortificante

dichiarazioni di voto)

Grazie,

Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, oggi, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, ho deciso di intervenire anche io in quest'Assemblea al fine di porre l'attenzione su un argomento che spesso viene sottaciuto, vale a dire le molestie e le violenze sessuali nelle Forze armate. L'uguaglianza, intesa come uguagliamento dei diversi, è un ideale permanente e perenne degli uomini viventi in società; ogni superamento di questa o quella discriminazione viene interpretata come una tappa del progresso civile: oggi più che mai, queste parole, pronunciate dal filosofo Noberto Bobbio, sono estremamente significative. Un rinnovamento della politica e soprattutto della società si realizza con il contributo congiunto e con una partecipazione sia delle donne, che degli uomini. L'ingresso del personale femminile nelle Forze armate, comprese Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, ha costituito un evento che nella coscienza comune è stato e forse viene ancora avvertito come la conquista da parte della donna di una nuova frontiera in una società che, purtroppo, è fortemente declinata al maschile.

a proporre norme di aggiornamento dei codici penali militari in tema di reati sessuali commessi da appartenenti alle Forze armate. Tale forte esortazione morale, prima ancora che politica, assume nuova portata e rilevanza nella giornata di oggi, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, con il forte auspicio che determini misure sempre più efficaci nel contrasto ai soprusi sessuali anche in ambito militare. L'ingresso della componente femminile nella compagine militare ha non soltanto comportato la necessità di adeguare le infrastrutture militari, ma anche imposto nel contempo un radicale cambiamento soprattutto nella mentalità. Il Ministro della difesa si è mostrato attento alla promozione e protezione dei diritti delle donne, ma, nonostante i tangibili progressi, da quando le donne sono entrate nelle Forze armate, nell'ordinamento militare non esiste una fattispecie autonoma di reato di violenza sessuale o molestia, essendo configurabile una semplice circostanza aggravante allorché il fatto sia commesso da un militare uomo. Per questi motivi, si rende necessario rafforzare gli strumenti giuridici di contrasto alle molestie e alla violenza sessuale mediante la prevenzione e la formazione, affinché si raggiunga la coesione e l'efficacia di tutti

Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero attirare la vostra attenzione sul sistema di accoglienza nelle comunità per minori e, in particolare, sugli episodi di violenza che si consumano soprattutto durante i turni notturni. Busto Arsizio: un'educatrice è stata aggredita da 4 minori in una comunità durante un turno di notte. Nuoro: 4 minorenni, ospiti di una comunità per recupero di minori con particolari disagi comportamentali, sono stati ritenuti responsabili di sequestro di persona, estorsione, violenza sessuale, *stalking*, maltrattamenti, lesioni e danneggiamento. Treviglio: un giovane viene arrestato per una violenza sessuale ai danni di un'educatrice durante il turno notturno. Bergamo: un giovane ospite della comunità una notte, dopo aver scassinato la porta della camera da letto dell'educatrice, si sarebbe introdotto furtivamente nella stanza mentre la giovane dormiva e avrebbe tentato di stuprarla.

Frosinone: un'educatrice è stata violentata e picchiata selvaggiamente da tre giovani che seguiva come *tutor* in una casa famiglia del Frusinate. Sono solo alcuni esempi degli episodi di violenza che si registrano nelle comunità di minori, soprattutto durante l'orario notturno. In molti casi si è scongiurato il dramma o l'episodio di violenza ha potuto trovare fine solo dopo l'intervento del collega che arrivava per il turno del mattino successivo. Sono solo esempi noti alla cronaca di persone che hanno avuto il coraggio di denunciare, laddove in molti casi si rinuncia a farlo, qualche volta - ahimè - anche perché scoraggiati dagli stessi gestori di queste strutture. Oggi 25 novembre, nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, io intervengo per chiedere a questa onorevole Assemblea di riflettere sulla necessità di intervenire con norme tecniche e contrattuali a tutela della figura dell'educatore, ad esempio prevedendo negli orari notturni un turno in compresenza che non lasci queste educatrici da sole dentro le comunità e dando maggiore dignità all'attività professionale svolta a servizio della comunità e dei giovani in particolari difficoltà.